Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, dopo l'intervento del rappresentante del Governo, ciascun Gruppo avrà a disposizione cinque minuti. Ha facoltà di parlare il ministro per i beni e le attività culturali, onorevole Bondi.

Onorevoli senatori,

Se invece vogliamo tutti far prevalere la serietà, l'obiettività e la misura, sarebbe giusto e corretto riconoscere che i problemi di Pompei si trascinano da decenni, come peraltro la situazione in cui versa l'intero patrimonio artistico italiano, senza che nessuno finora sia riuscito a risolverli e ad impostare una strategia efficace. Sarebbe comodo addossare a me tutte le responsabilità, oppure addossarle al Governo, accusato di tagliare i fondi alla cultura.

Bisognerebbe anche avere il senso della misura ed evitare ogni strumentalizzazione politica. Vi sono stati negli ultimi anni altri crolli, della stessa gravità, se non più gravi ancora, in altre aree archeologiche del nostro Paese. Nell'aprile del 2001, ad esempio, è crollato un tratto delle Mura aureliane,

a nessuno - giustamente - è venuto in mente di chiedere le dimissioni del ministro Melandri. Se nel mio caso valgono altri criteri, ne prendo atto. Chiedete pure le mie dimissioni; ricorrete addirittura ad una mozione di sfiducia personale. Ma se devo saltare su una mina, come ha detto l'onorevole Franceschini, per far esplodere le contraddizioni di questa maggioranza, allora è un altro discorso, che non c'entra niente né con la cultura né con Pompei. *(Applausi La cosa che mi rattrista di più non è di subire un trattamento così ingiusto e pretestuoso, perfino violento, nei confronti della mia persona, ma di vedere a quali livelli di incattivimento e di meschinità è giunta la vita politica italiana.

un grande lavoro, che ha dato alcuni primi risultati importanti. Qualcuno ricorda in quest'Aula le condizioni in cui si trovava due anni fa l'area archeologica di Pompei? La stampa aveva denunciato una situazione incredibile ed intollerabile per l'immagine dell'Italia: sporcizia ovunque, mancanza di servizi igienici, cani randagi, guide non autorizzate che intimidivano in alcuni casi i turisti stranieri, ristoranti abusivi, *domus* chiuse al pubblico da decenni. Questa era la situazione in cui si trovava Pompei due anni fa. Sulla base di questa situazione di emergenza ho deciso di nominare un commissario, anche perché i soprintendenti mi avevano fatto capire di essere inadeguati ed impossibilitati ad affrontare alcune questioni che riguardavano l'ordine pubblico in un territorio complesso e delicato com'è quello campano, e quello di Pompei in particolare.

a verificare di persona quello che è stato fatto in questi due anni: vi rendereste conto di quali progressi abbiamo fatto in due anni di lavoro La decisione di nominare un commissario, onorevoli senatori, nasceva certamente dall'emergenza, ma anche dalla mia convinzione che un'area archeologica vasta, immensa, complessa come Pompei, una delle aree archeologiche più importanti

c'è una cattiva informazione a questo riguardo), il commissario ha lavorato sempre in stretto raccordo e in totale sintonia con i soprintendenti e ha operato solo sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni degli stessi: il il commissario è stato il braccio operativo, in qualche modo, dei soprintendenti. Nei due anni di commissariamento, dal giugno 2008 al giugno 2010, giorno in cui è cessato il commissariamento per tornare alla normalità, sono stati investiti oltre 79 milioni di euro, dei quali 21 milioni provenienti dai fondi FAS del Ministero dello sviluppo economico, 40 milioni dai residui attivi giacenti nel bilancio della soprintendenza speciale di Napoli e di Pompei e 18 milioni derivanti dalla vendita dei biglietti. Di questi fondi, l'83 per cento è stato destinato alla messa in sicurezza dell'area archeologica (per un ammontare di 65 milioni di euro), consentendo la manutenzione, il restauro e l'apertura al pubblico di un numero considerevole di edifici. In seguito a questo lavoro, infatti, è stato possibile aprire per la prima volta al pubblico 49 edifici monumentali (nel 2008 ne erano aperti soltanto 37) aperti soltanto 37) e 23 *domus* (nel 2008 ne erano aperte soltanto 11). Nelle prossime settimane, inoltre, verranno avviati i lavori che riguardano altre cinque importanti *domus*, tra cui la celebre Villa dei misteri. È doveroso ricordare altri risultati ottenuti dalla gestione commissariale: l'apertura di un primo soccorso dentro gli scavi, che non c'era, e una convenzione con la Croce Rossa Italiana per la sua gestione; una nuova organizzazione del servizio delle guide turistiche (prima il servizio era quasi totalmente in mano all'abusivismo e lavoravano meno di 20 guide, che esercitavano un'attività di intimidazione sulle altre, mentre oggi sono iscritte più di 200 guide, tutte regolari, tra cui tante donne e giovani);

il recupero della legalità in molti settori, attraverso una collaborazione con le forze dell'ordine, la prefettura e la questura di Napoli; il contrasto all'abusivismo commerciale, dentro e fuori l'area archeologica; una campagna di lotta al randagismo, condotta in collaborazione con le associazioni animaliste; una nuova sede della soprintendenza, che era ancora nel *container* dopo il terremoto del 1980. Anche grazie a questo lavoro, nel 2010 c'è stato un aumento del 40 per cento del turismo scolastico e un aumento medio di circa il 15 per cento dei visitatori e degli incassi. Il crollo di un edificio, per quanto grave sia, e per quanto grande sia il valore simbolico di questo fatto (che io non ignoro, proprio per il valore simbolico che l'area archeologica di Pompei

in realtà a Pompei è avvenuto il crollo di ciò che era stato restaurato negli anni '50, perché l'edificio sottostante, compresi gli affreschi, è rimasto - per fortuna

Perché è avvenuto il crollo? A giudizio della soprintendenza, nessun elemento faceva presagire il crollo dell'edificio, anche se le forti piogge avevano causato qualche giorno prima un piccolo cedimento nel vicolo adiacente. Chi pensa veramente che un'area archeologica che un'area archeologica come Pompei, con 1.500 edifici che risalgono a più di 2.000 anni fa, possa essere immune da problemi e cedimenti è una persona che non ha il minimo senso della realtà. Un sopralluogo, effettuato venerdì 5 novembre da parte dell'ufficio tecnico, non aveva segnalato pericoli visibili per la *schola*. Da quanto è stato possibile rilevare fin dal primo sopralluogo effettuato dalla soprintendenza dopo il crollo, la copertura in cemento armato dell'edificio - che come ho ricordato fu realizzata con i restauri del dopoguerra - è collassata, cadendo in gran parte all'interno dell'edificio, provocando soltanto il crollo della parte superiore e delle mura perimetrali della facciata. Verosimilmente - ma si tratta di accertamenti ancora in corso - il crollo ha interessato le murature verticali, ricostruite nel dopoguerra, e la copertura, mentre parrebbe essersi conservata la parte più bassa di quelle medesime parti, e cioè la parte che ospita le decorazioni affrescate, che quindi si ritiene potrebbero essere recuperate. Sulla copertura in cemento armato era stato recentemente eseguito un lavoro di manutenzione per l'impermeabilizzazione, pertanto si esclude che il danno sia da mettere in relazione ad infiltrazioni nel solaio che ne abbiano minato la tenuta. Allo stato dei primi accertamenti, il dissesto che ha provocato il crollo sembrerebbe imputabile alla pressione sviluppata sulle murature perimetrali dal terrapieno che si trova a ridosso della costruzione e che, per effetto delle abbondanti piogge di questi giorni, doveva essere completamente imbevuto di acqua. Alla luce di queste condizioni, che interessano altri edifici, purtroppo non si possono escludere altri cedimenti (naturalmente perché vi sono altri edifici che si trovano a ridosso del terrapieno costituito dalle aree ancora da scavare, e che rappresentano ancora un terzo dell'antica città di Pompei. Onorevoli senatori, poiché il Presidente della Repubblica ha chiesto, giustamente, che qualcuno dia delle spiegazioni e lo faccia senza ipocrisie, non mi sottrarrò a tale obbligo. Lo farò: sto offrendo delle spiegazioni, senza ipocrisie, e soprattutto senza scaricare le responsabilità su altri e, ancor meno, sulla mancanza di fondi. Onorevoli colleghi, la mancanza di fondi - voglio dirlo chiaramente - almeno per quanto riguarda Pompei non è assolutamente la causa di ciò che è accaduto. Sarebbe comodo da parte mia dirlo. Se dicessi che tutto è accaduto per mancanza di fondi potrei perfino accampare meriti come paladino della cultura contro i tagli del Governo.

nel 2005, a 75 milioni di euro; nel 2006, a 48 milioni di euro; nel 2007 a 49 milioni di euro; nel 2008, a 43 milioni di euro; nel 2009, a 25 milioni di euro; nel 2010, fino ad ottobre, a 27 milioni di euro. Questi dati, onorevoli senatori, dimostrano che il problema vero non è la mancanza di fondi,

il nostro patrimonio storico-artistico e il nostro paesaggio, questo lo si deve in gran parte al lavoro che hanno svolto i nostri soprintendenti.

dovrebbe essere quella di garantire, come hanno fatto fin qui, la tutela del nostro patrimonio storico-artistico. La mia opinione è che l'unico modo per affrontare alla radice il problema di Pompei di lasciare ai soprintendenti il compito della tutela, mentre quello della gestione e dell'applicazione dei progetti di manutenzione e di restauro, predisposti dagli stessi soprintendenti, debba essere assegnato a nuove figure professionali e secondo nuove forme di gestione. Per questo, l'ufficio legislativo del Ministero sta predisponendo le linee operative per la definizione degli atti costitutivi e statutari di una fondazione per la gestione di Pompei, come è stato proposto di recente anche dall'ex ministro per i beni e le attività culturali, senatore Rutelli. Soprintendenti e *manager* dei beni culturali, che vengono formati dalle nostre università e che restano senza lavoro, devono collaborare insieme: restano senza lavoro, devono collaborare insieme: questa, secondo me, è la soluzione. Per questo, ho costituito qualche giorno fa un gruppo di lavoro, coordinato dal professor Carandini, presidente del Consiglio nazionale dei beni culturali nonché uno dei più autorevoli archeologi italiani, di fama internazionale, e formato dal dottor Cecchi, segretario generale del Ministero, dal professor De Caro e dal professor Proietti, allo scopo di formare un gruppo di studiosi che valuti innanzitutto lo stato di degrado e il livello di rischio di tutti gli edifici dell'area archeologica di Pompei, che rilevi attraverso le moderne tecnologie l'intera città per preservarne la documentazione e che prosegua l'opera di studio e di catalogazione di tutti gli edifici. Questo gruppo di lavoro dovrà affiancare d'ora in avanti la soprintendenza e dettare le linee di intervento e le priorità.

Per far fronte alle emergenze in tutto il Paese, oggi sarebbe necessario autorizzare l'assunzione di almeno 50 architetti e di almeno 80 archeologi.

se volete addebitarlo a me, fatelo pure, ma - lo ripeto - ha una lunga storia, che secondo me nasce da una sottovalutazione, non di questo o di quel Governo, bensì da una sottovalutazione che le classi dirigenti

Sono presenti in tribuna una delegazione dell'Istituto di istruzione superiore statale «John von Neumann» ed una delegazione della Confraternita dell'Università di Heidelberg (Germania). Ad esse rivolgiamo il saluto dell'Assemblea.

La causa immediata più probabile sono state le perduranti condizioni di maltempo, mentre le cause di fondo sono verosimilmente il peso di un restauro in cemento armato realizzato all'inizio degli anni '50, e presumibilmente non appropriato, ma soprattutto la mancanza di controllo e di manutenzione. La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo,

La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo, creando enorme imbarazzo al nostro Paese, la cui immagine è risultata inequivocabilmente danneggiata. l'aspetto peggiore, ovviamente (e questo non lo dobbiamo dimenticare), è la perdita di un pezzo importante del nostro patrimonio culturale, quel patrimonio che noi abbiamo la responsabilità di preservare e trasmettere indenne alle generazioni future. Questo è il punto più rilevante, perché la conservazione del patrimonio culturale è uno degli aspetti più importanti

infatti, che il legame con il territorio si affievolisce, fino a scomparire. E questo si traduce poi nell'incuria, che porta al dissesto idrogeologico, causa prima dei danni di questi giorni. Dinanzi a questo avvenimento, tutti hanno richiesto un accertamento delle responsabilità ai vari livelli, e prioritariamente una precisa assunzione di responsabilità da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali. A questo proposito, ci associamo innanzitutto alla generale richiesta di accertamento delle responsabilità in capo alle figure tecniche e istituzionali coinvolte a tutti i livelli,

di una chiara iniziativa nei riguardi della politica del Governo: una politica di continui tagli di risorse al bilancio del Ministero, nonostante la situazione di evidente e generalizzata emergenza che investe i beni culturali in tutto il Paese, in tutti i settori, e non solo nel sito di Pompei. Dinanzi a questa politica, e nei confronti di chi sottolinea la subalternità della cultura ad altri obiettivi per giustificare gli ingenti e ripetuti tagli di risorse, ci saremmo aspettati dal Ministro una proposta di cambiamento radicale di rotta nella gestione del patrimonio culturale italiano: una nuova impostazione che facesse meno ricorso alle normative d'emergenza, curasse di più e con più attenzione l'ordinaria manutenzione e quindi pretendesse adeguati stanziamenti di risorse. Abbiamo udito sempre più spesso negli ultimi anni la parola «valorizzazione» del patrimonio culturale italiano. E questa parola quasi sempre è associata, giustamente, al sostegno e al rilancio del settore turistico, importante per la nostra economia.

per assicurare la sopravvivenza della risorsa principale da valorizzare, cioè il patrimonio. Ma se è così, allora, abbiamo confuso la parola «valorizzazione» con ciò che è invece una pura e semplice speculazione. Forse è il caso di prendere coscienza che il nostro enorme patrimonio artistico e culturale ha bisogno di meno operazioni di *marketing* e di più risorse per la manutenzione e la conservazione, perché solo così potremo assicurare la sua sopravvivenza a beneficio delle future generazioni. Questa, infatti, voglio ripeterlo, è la nostra vera e principale responsabilità. Ci riserviamo ovviamente di proporre attraverso gli idonei atti parlamentari le iniziative opportune a tutela del patrimonio culturale della Campania e dell'Italia.

i dettagliati ma inutili resoconti di quanto accaduto in questa povera Italia stanno imperversando in quest'Aula da ormai troppe sedute. Ieri si discuteva dell'Italia sotto l'acqua e sulle possibili cause. L'altro ieri è stata la volta del ministro Maroni che troppo frettolosamente ha definito chiuso il caso Ruby ma che, stando alle dichiarazioni del pubblico ministero che si occupò della faccenda, chiuso non è. Oggi siamo qui a discutere sulla *domus* dei gladiatori, così ingloriosamente venuta alla ribalta. Un'Italia che, per raccontarla per capitoli, è sotto l'acqua. E a proposito, quale potente ministro del Sud accompagnerà il *Premier* a verificare gli ingenti danni provocati nel Cilento dal maltempo? O saranno usati anche questa volta due pesi e due misure a scapito delle Regioni meridionali? ancora sotto l'immondizia, e mi chiedo che fine ha fatto il miracolo di due anni fa. Era un vero miracolo o era soltanto un po' di spazzatura buttata sotto il tappeto? Ed è anche un'Italia sotto i crolli, che non sono solo materiali ma anche e soprattutto etici e morali. Signor Ministro, vuole che a confutazione della sua informativa le legga quello che sul caso hanno detto e scritto autorevoli esperti, come il professor Settis ed altri? Vuole che le ricordi, come hanno fatto e faranno altri autorevoli colleghi, gli innumerevoli episodi accaduti sotto la sua gestione, come il crollo nella Casa dei casti amanti, la caduta di un pezzo del Colosseo, la frana della volta della *Domus aurea*?

Ma ad onor del vero, penso che qui manchi il «convitato di pietra». Manca in quest'Aula il vero responsabile di quello che sta accadendo. Manca, non come si ostina a dire qualcuno, il fato, ma il ministro Tremonti, che con i suoi famigerati tagli lineari ha indebolito la qualità degli interventi di cui un patrimonio come quello posseduto dal nostro Paese aveva ed ha bisogno. Ebbene, a me hanno insegnato che in tempo di vacche magre tra un ridimensionamento delle spese per le vacanze o delle spese per la cultura non ci debbano essere perplessità: si rinviano le prime e si implementano le seconde. Così non è stato. Onorevole Ministro, *quisque faber fortunae e la sua buona volontà, le buone intenzioni cozzano con l'amara realtà. Signor Ministro, io penso che le dimissioni che le sono state chieste non le si debbano chiedere e che lei debba lasciare, *sua sponte*, per non essere riuscito ad ottenere i fondi necessari per il suo Ministero. Ma noi dovremmo invece chiedere le dimissioni del ministro Tremonti e del suo Governo che ha avallato tali scellerate scelte. E le voglio dire, a conclusione,

ha ripetuto ancora una volta che il crollo della *domus* dei gladiatori è stato - e questa è la sua unica linea difensiva una non sua responsabilità e ha detto testualmente: «Se avessi responsabilità per ciò che è accaduto sarebbe giusto chiedere le mie dimissioni, anzi le avrei date io». Poi ha ancora detto: «Se invece facciamo prevalere serietà, obiettività e misura, allora sarebbe giusto riconoscere che i problemi di Pompei come le situazioni in cui versa il patrimonio artistico si trascinano da decenni, senza che nessuno sia riuscito a risolverli definitivamente». Vede, signor Ministro, io credo che quando un uomo di Governo afferma che tutti hanno responsabilità in questa o in quella tragedia - ed è quello che lei ha fatto ieri, sta facendo da molti giorni e ha fatto ancora oggi - è chiaro che ci troviamo di fronte al solito tentativo, di indimenticabile ideazione craxiana, del «siamo tutti ladri, quindi nessuno è ladro». Signor Ministro, io non credo che questa sua difesa sia accettabile; responsabilità esistono, per il passato, per il presente e per il futuro. E allora veniamo al presente e al recente passato, che sicuramente la riguarda e che è frutto delle decisioni del Dicastero di cui lei ha la responsabilità. Per essere espliciti, sto parlando di una cosa molto precisa: l'ingresso della Protezione civile a Pompei. In sostanza, il Governo Berlusconi aveva equiparato la situazione di Pompei a un'emergenza tale (addirittura immaginando che ci potesse essere un imminente rischio di eruzione del Vesuvio), da richiedere l'incarico al Dipartimento di Bertolaso e, quindi, in questo modo, da consentire di agire in deroga alle norme e, soprattutto, di evitare il controllo preventivo delle delibere: insomma, agire con mano libera. Oggi abbiamo appreso, signor Ministro, dalle sue parole che questa urgenza era sostanzialmente per rifare e riaprire i bagni pubblici. La Corte dei conti - lei lo sa, signor Ministro - ha pubblici. La Corte dei conti - lei lo sa, signor Ministro - ha sonoramente bocciato l'ingresso della Protezione civile a Pompei. La magistratura contabile ha ribadito che il Dipartimento della protezione civile può svolgere non qualsiasi attività, ma «l'attività finalizzata alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali(...), che determinino situazioni di grave rischio». La Corte le ha contestato, signor Ministro, l'esclusione dai controlli delle decisioni che, per esempio, riguardano «le opere di manutenzione straordinaria per consentire la piena fruizione dei beni archeologici» o «l'organizzazione dei servizi di guida ai turisti» o le modalità di sponsorizzazione ma alla fine in un certo senso, la Corte è stata con amarezza costretta ad arrendersi. Sempre la Corte nel suo provvedimento, dice che non può ignorarsi che, di fatto, tutti i provvedimenti, di cui è stata chiesta (inutilmente) la trasmissione al controllo preventivo di legittimità, hanno già esaurito la loro operatività. In un esposto presentato da una forza sindacale è stato rilevato che in un affidamento per il restauro e la sistemazione del complesso dei teatri negli scavi la ditta era RTI Caccavo con una spesa molto ingente, e nel 2010, dopo pochi mesi, veniva sottoscritto un altro affidamento per opere complementari, e la ditta era sempre la stessa, pur mancando qualsiasi parere del comitato tecnico‑scientifico per i beni archeologici. E che dire poi della mostra «Pompei e il Vesuvio. Scienza, conoscenza ed esperienza», affidata alla società Comunicare Organizzando, la stessa che gestisce le mostre allestite per il G8 nella caserma di Coppito?

con una previsione per il 2011 e il 2012 che passerà da 21 a 15 milioni di euro: se non sono tagli questi, non so come li vogliamo chiamare! Ma anche ammesso che lei abbia ragione, e che quindi le risorse siano sufficienti ma vengano mal gestite, allora, Ministro, mi pare che lei renda una dichiarazione confessoria delle sue colpe, perché i fatti ci dimostrano - ed è ancora peggio - che le risorse non sono state per nulla ben gestite. L'ultimo punto su cui la voglio far riflettere è il tema della soprintendenza di Napoli e Pompei che ormai da troppo tempo è senza una guida strutturale. A settembre, signor Ministro, dopo la pubblicazione del bando, sembrava certa la nomina del nuovo soprintendente, ma agli inizi di ottobre, senza spiegazioni, il bando è stato annullato. Si è detto che un altro bando sarebbe stato fatto nel mese di novembre. Intanto, Pompei non poteva rimanere senza un responsabile. Quindi è stato affidato un nuovo *interim* fino a dicembre. Adesso il cuore del problema è nel futuro di questo luogo straordinario, che è anche la più importante impresa economica dell'area. Nel 1997 - lo ricordo all'Assemblea anche se tutti lo sappiamo - l'UNESCO ha dichiarato Pompei patrimonio mondiale dell'umanità. Quindi è chiaro che è per noi una risorsa importantissima. Non c'è equivalente in nessuna altra parte del mondo. Bene, signor Ministro, stiamo all'11 novembre e del bando per il nuovo soprintendente non c'è traccia. Non abbiamo ascoltato dalle sue parole un'idea complessiva della futura gestione di Pompei che sia credibile e accettabile. Allora forse, signor Ministro (mi permetta, con tutto il rispetto che le devo), anche per meglio poter occupare il suo tempo nelle inutili quanto oziose difese del *Premier* per il caso Ruby, dovrebbe dimettersi, e l'Italia dei Valori chiede a lei e a tutto il Governo di dimettersi.

il crollo dell'Armeria del gladiatore, così come ha detto giustamente il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, è una vera vergogna nazionale. E questo lo è a prescindere - lo dico subito da eventuali responsabilità politiche, istituzionali e amministrative, perché il danno di immagine che nel mondo questa vicenda ha ha determinato, diretto o indiretto, anche dal punto di vista patrimoniale, rispetto alla capacità attrattiva di quel sito, che è sottoutilizzato ma che sempre attrattivo è, è tale che deve indurre tutti noi a fare una riflessione impietosa sullo stato di questo Paese, a prescindere dalle questioni di carattere politico che ci interessano, e parecchio, come dirò, ma che in questo momento recedono rispetto alla vicenda di Pompei. Voglio dire questo, signor Ministro, perché proprio per questa ragione avremmo apprezzato di più un'analisi più chiara sulla vicenda delle cause che hanno riguardato il crollo dell'Armeria. Infatti, sinceramente dalle sue parole non abbiamo compreso

un intero villaggio, come è successo un anno fa a Giampilieri con 33 morti, o un'intera Regione si blocca e blocca il suo processo produttivo ed economico (mi riferisco al Veneto). L'Armeria dei gladiatori gladiatori collassa. Se è una tragica fatalità non lo so, ma certamente a queste tragiche fatalità - che ormai hanno una frequenza tale

di un problema che riguarda incapacità di natura amministrativa, tecnica e gestionale. Mi associo alle sue parole nei confronti dei soprintendenti. Devo dire che lei, con onestà, ha fatto qui oggi un'affermazione che non le ho sentito fare, per la verità, alla Camera, cioè

Questo lo afferma anche il segretario generale del suo Ministero, quando riferisce che in questo Paese non si fa manutenzione ordinaria dei beni culturali da 50 anni. D'altro canto, anche il sindaco di Pompei non è stato tenero rispetto a questa vicenda, affermando che si trattava e si tratta di una vicenda obiettivamente prevedibile. Se si tratta, signor Ministro, di una questione di carattere amministrativo, io credo che l'attività di accertamento delle responsabilità debba essere impietosa, perché la formula della gestione straordinaria attraverso il sistema "sperimentato" della Protezione civile, con la nomina di un commissario straordinario per l'area archeologica di Pompei, è un sistema che ha fallito. Infatti, proprio con la nomina del commissario, che lei ha rivendicato come merito di questo Governo e che doveva servire a realizzare alcuni interventi (che sono stati doveva dotare l'area di strutture che fossero nelle condizioni di avere un controllo capillare del territorio dell'area archeologica, prevedendo che se piove e se un terrapieno è se vi è un solaio realizzato in cemento armato, per tecniche di restauro risalenti agli anni '50, è assolutamente prevedibile (per chi non fa questo mestiere: figuriamoci per chi lo fa) che quella struttura possa, e anzi debba, collassare. Da questo punto di vista, le dico con grande serenità e sincerità che le sue parole non ci hanno rassicurato ma, in qualche modo, ci hanno preoccupato ulteriormente e sconcertato. Infatti, se il problema non è rappresentato dalle risorse per l'area archeologica di Pompei, ma vi è una incapacità delle strutture tecniche e amministrative di gestire quel sito archeologico, io ritengo che, poiché dopo tre anni di attività, comunque, tali fatti sono noti e si correggono, una responsabilità ci sia e che essa debba essere accertata senza se e senza ma, da ogni punto di vista.

ma constatiamo un fatto molto grave: nella manovra finanziaria per il 2011 è previsto, proprio alla voce tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistiche, un taglio di oltre 200 milioni di euro. Questo è un fatto politico di enorme portata, soprattutto alla luce della gravità della vicenda che ha riguardato Pompei e che, come da lei affermato in quest'Aula, si può ripetere, e rispetto alla quale lei manifesta un'impotenza da parte del Ministero e delle strutture competenti a far fronte a questo tipo di situazione.

parole di maggiore determinazione, soprattutto nel rapporto e nell'attività che questo Governo deve svolgere in questo settore. Non bastano i gruppi di studiosi. Essi sono importanti, ma anche questa sembra una toppa rispetto al buco, alla voragine che si è creata.

ma in ogni settore, non serve più la politica degli *spot* e degli effetti speciali, che servono solo a rinfrescare l'immagine ma non incidono sul contenuto e sulla sostanza dei problemi. Infatti, se in questo Paese, contemporaneamente, il Nord si blocca per un'alluvione, così come si blocca anche il Sud per le alluvioni costanti, se la Campania è ancora prigioniera della spazzatura, se crolla l'Armeria di Pompei, ciò significa che c'è una cultura dell'amministrazione, che è politica e amministrativa, che certamente non riguarda solo il suo periodo di gestione (ma noi oggi di quello parliamo), che è al capolinea e che ha prodotto in questi anni tante chiacchiere, ma non ha prodotto alcun effetto positivo rispetto ai problemi strutturali di questo Paese. Perché noi diciamo che Pompei è una metafora? Non perché vogliamo attribuire una responsabilità personale su questa vicenda, ma perché la questione di Pompei, come tutte le altri questioni riguardanti, ad esempio, il sistema infrastrutturale del nostro Paese, è stata coltivata con la logica del consenso elettorale immediato e non nella logica della cultura dell'ordinaria amministrazione, che è quella che salvaguarda il paesaggio, l'ambiente e i siti archeologici. Oggi la spettacolarizzazione della politica è arrivata a livelli indecenti insopportabili, che stanno facendo crollare il sistema, perché le istituzioni non sono nelle condizioni di dare risposte, e certamente non sono risposte che si danno nel breve periodo. Dopo sedici anni di bipolarismo, mi faccia dire, è chiaro che, nel momento in cui non si fanno scelte che siano impopolari o di medio e lungo periodo, ma solo scelte che servono a vincere questa o quella campagna elettorale, il risultato è la spazzatura di Napoli, il crollo dell'Armeria di Pompei, l'alluvione nel Veneto, con buona pace del federalismo di bottega;

crolla la Scuola dei gladiatori di Pompei ed è scandalo. Le opposizioni chiedono le dimissioni del Ministro dei beni culturali, ma per loro l'importante non sembra tanto scoprire le dimensioni del danno, e men che meno capire il perché una cosa del genere sia potuta accadere. Per la stampa progressista ciò che conta è coprire di fango il Ministro, raccontando che non ha contribuito adeguatamente alla manutenzione degli scavi, sostenere che a causa dell'incuria del centrodestra uno splendido monumento è rovinato. Cosa, guarda caso, non successa quando si verificarono i primi crolli della *Domus aurea* (ministro Giovanna Melandri, della sinistra), o ancora il crollo, straordinariamente grave, di un lungo tratto delle Mura aureliane, che vennero giù a Porta Ardeatina, crollo di pertinenza del Comune di Roma ma sotto la tutela del Ministero (a guida progressista), di cui parlò tutto il mondo e che il centrodestra non strumentalizzò, dimostrandosi più cauto e responsabile. La sinistra, al contrario, si gioca l'ultimo filo di credibilità cercando di far passare il messaggio che a Pompei siano state tolte le risorse per gestire un patrimonio archeologico tanto importante, facendo finta di non sapere che la soprintendenza di Pompei incassa più di quanto spende: ogni anno circa 22 milioni di euro, di cui 8 impiegati per i restauri. Non sono i soldi che mancano. Con Rocco Buttiglione ministro dei beni culturali, si accumularono nelle casse della soprintendenza 30 milioni di euro. Gli scavi di Pompei sono stati commissariati nel giugno 2008, dopo che i mezzi d'informazione ne avevano denunciato lo stato di degrado: scavi chiusi per assemblee sindacali improvvisate dai custodi, guide abusive, addirittura un ristorante abusivo presente all'interno degli scavi, assenza di protezioni sanitarie. Di comune accordo con la Regione Campania (governata dal centrosinistra), il Governo decise il commissariamento. Cosa però che non esautora la soprintendenza di Pompei: il commissario deve lavorare in accordo con il soprintendente e tutti gli interventi sono vincolati all'intesa con quest'ultimo. Tra luglio 2008 e giugno 2010 i commissari hanno mobilitato risorse per 79 milioni di euro, di cui circa 65 per la messa in sicurezza di varie aree, e fra gli interventi urgenti - di cui era stata richiesta la mappatura - nessuno ha segnalato la Scuola dei gladiatori. Dove sta la colpa del Ministro? C'è poi da più parti l'accostamento improprio tra gli smottamenti al Sud e le tracimazioni al Nord. Da una parte, però, spesso grandi risorse sono state impiegate male, dall'altra le risorse sono state tolte, impedendo una buona gestione del territorio. Subire le conseguenze di abusivismo e disordine non è come dover affrontare uno sviluppo abnorme senza poter disporre di adeguati strumenti economici. In questi giorni assistiamo al disastro del Veneto: 50 centimetri di acqua caduti solo in pianura (durante l'alluvione del 1966 furono 20 centimetri); 121 Comuni colpiti; 5.000 aziende agricole messe al tappeto; 3.000 attività produttive che hanno subito danneggiamenti o disagi a causa del diluvio; 10.000 ettari di terreno sott'acqua. Il residuo fiscale del Veneto (la differenza cioè tra quanto i cittadini versano allo Stato tra tasse, imposte e contributi previdenziali e quanto rientra in termini di trasferimenti al territorio) è di quasi 5 miliardi di euro l'anno: è la cifra della solidarietà veneta nei confronti delle altre Regioni. Comprensibilmente ora chiedono di avere indietro almeno una parte di questi soldi per affrontare l'emergenza, ma pure questa richiesta è stata utilizzata dalla sinistra per gettare fango sugli avversari politici. Quando si è sparsa la voce che dopo il crollo della Scuola dei gladiatori qualcuno era già pronto a chiedere fondi per Pompei, Luca Zaia, governatore del Veneto, è giustamente sbottato affermando che i soldi andavano dati prima agli alluvionati, poi a Pompei e dicendo: «Abbiamo mezzo milione di persone sott'acqua», battuta puntualmente e vigliaccamente strumentalizzata dalla sinistra per richiamare l'immagine, cara a quella parte, del leghista rozzo e ignorante. anche in questo caso, di recuperare consensi sfruttando le disgrazie per colpire l'avversario politico? Dubitiamo che i cittadini siano tanto sprovveduti.

tra tutte le cariche pubbliche del nostro Paese quella più invidiata è certamente proprio la sua: quella di Ministro dei beni culturali. Il suo è un Ministero difficile, ma molto bello. Le è stata affidata la ricchezza più preziosa del nostro Paese; una ricchezza di fascino straordinario e di fama mondiale, che non ha soltanto un immenso valore economico e che non è solo il motore del nostro turismo: nei beni culturali noi troviamo le nostre radici, la nostra identità culturale. È nei beni culturali che c'è il nostro essere una grande Nazione con una grande storia. Signor ministro Bondi, le faccio notare il vuoto

Non sarà, signor Ministro, che anche nella sua maggioranza si sono accorti *(Commenti del senatore Monti)* che lei non è stato all'altezza del patrimonio che le è stato affidato e che ora, con il crollo a Pompei della Casa dei gladiatori, vengono alla luce i suoi gravi errori gestionali, ordinamentali e politici? Temo che, scegliendo lei, il presidente Berlusconi non si sia preoccupato della sua attitudine a fare il Ministro, quanto - con la nota mancanza di senso dello Stato che gli è propria - della sua fedeltà, che per lui conta più di qualsiasi competenza ministeriale. Sono altre le sedi in cui verrà valutato se e per quanta parte il crollo della Casa dei gladiatori è dovuto all'incuria e alla colpa. la sua idilliaca ricostruzione di poco fa dimostra una plateale sottovalutazione del rischio da parte del Ministro dei beni culturali. In Senato noi dobbiamo considerare le sue responsabilità politiche, se ci sono, ma dobbiamo cominciare da questa inaccettabile e - mi permetta - troppo svelta autoassoluzione con la quale lei si è tirato fuori dalle sue responsabilità. Il suo primo errore, signor Ministro, è quello di essersi messo sul solco di Berlusconi nell'utilizzo delle ordinanze di Protezione civile per la gestione dei più delicati siti archeologici del nostro Paese, da Pompei all'area archeologica di Roma, Foro romano compreso. Queste sono scelte sue, sono scelte politiche, che hanno sottratto il potere d'intervento agli archeologi, per attribuirlo a dirigenti della Protezione civile.

al di là di ogni valutazione sulle persone, è proprio l'impianto ordinamentale ad essere sbagliato; e non lo diciamo adesso, a disastro avvenuto: lo abbiamo già denunciato già più volte qui nell'Aula del Senato. più volte esposta pubblicamente dal presidente Berlusconi, l'Italia deve essere governata con decreti-legge e ordinanze di Protezione civile, e Berlusconi lo ha fatto, con tanto di affidamenti diretti e di personale impiegato senza concorsi pubblici. Signor Ministro, il suo errore è stato proprio questo: l'essersi sollecitamente accodato - forse per fedeltà, forse per incapacità - alla disinvoltura con la quale Berlusconi ha governato l'Italia, senza riflettere sul fatto che Pompei e il Foro romano sono cose molte diverse dalle alluvioni e dai terremoti, e non sono neanche dei grandi eventi. L'altro suo gravissimo errore, signor Ministro, è stato non aver saputo o voluto fare del nostro patrimonio culturale una priorità assoluta tra le politiche del Governo;

sia stato il suo impegno a difesa del suo Ministero. Lei non è solo il Ministro dei beni culturali: è anche coordinatore del partito di maggioranza. Lei è nel cuore del presidente Berlusconi; lei è un uomo politico molto influente, e forse, per questo, avrebbe dovuto già dimettersi da tempo, per essere così potente nel suo partito, ma così fallimentare nella difesa dei beni culturali del suo Paese. *(Applausi dal Gruppo* *PD)*. L'Italia brucia ogni anno 70-80 miliardi di interessi sul debito - che Berlusconi ha portato dal 104 al 118 per cento del PIL - e rinuncia ogni anno a 100-150 miliardi di evasione fiscale. Nessun Paese in queste condizioni è in grado di sostenere una vera politica economica fatta di grandi decisioni e grandi investimenti pubblici. Ma anche gli Stati, come le persone, signor Ministro, quando le risorse sono limitate debbono saper scegliere come impiegarle al meglio e non buttarle via in scelte capricciose. lei ha colpevolmente taciuto quando il suo Governo sperperava e non ha difeso il suo Ministero. Lo ha detto anche lei in tempi passati, arrivando anche ad annunciare che forse si sarebbe dimesso. Non credo alla sua versione di poco fa, che i fondi non mancano e che le responsabilità sono della gestione, perché, se così fosse, le sue colpe sarebbero immense, dal momento che la gestione è cosa sua. Lei è Ministro da due anni e mezzo: di che cosa si è occupato, se non della gestione del suo Ministero e delle soprintendenze? *(Applausi dal

in Parlamento. Poco fa lei ha ricordato che l'Italia ha il record negativo di investimenti pubblici in cultura: ma noi non l'abbiamo mai sentita dimettersi, né votare contro quando venivano gettati al vento 3 miliardi per privatizzare l'Alitalia, che oggi Air France si appresta ad acquisire gratis. *(Applausi dal Gruppo* *PD)*. Pensi a quanta prevenzione si sarebbe potuta fare con quei 3 miliardi!

Perché non si è dimesso o non si è dissociato, votando contro, quando si è accorto di questo fiume di denaro che si spandeva ovunque, ma non arrivava mai là dove si difendono i nostri beni culturali?

ha stanziato 12 miliardi per istruzione, ricerca e sviluppo, oltre a 1,5 miliardi per la cultura. Finanziando la cultura, questi Paesi investono nel loro futuro e non buttano via i soldi solo per il gusto di poter dire d'aver promosso una cordata di volenterosi per l'Alitalia. La sua più grande La sua più grande responsabilità politica, signor Ministro, è stata quella di essere complice di un uomo che di Pompei non sa nulla e che quando si parla di cultura pensa subito alla televisione e al «Grande fratello». È per questo fallimento generale che lei deve dimettersi, per la *débâcle* della tutela, per lo sciopero di domani di tutti i musei italiani, per la crisi del teatro e per la difficoltà del cinema italiano.

che gli italiani sappiano apprezzare chi si assume con dignità le proprie responsabilità. Vorrà dire che lei se ne andrà tra non molto, quando non lei ma Berlusconi salirà al Quirinale a presentare le sue dimissioni al Capo dello Stato; ed in fondo, debbo dirle, è anche giusto, perché Berlusconi è responsabile almeno quanto lei, ministro Bondi, del crollo della Casa dei gladiatori.

sembra che nessuno abbia avuto modo o voglia di ascoltare quello che è stato detto dal ministro Bondi nel suo intervento. È così che noi abbiamo sentito giudicare il suo discorso, in ultimo dal senatore Zanda, che ha mescolato tutto in un'insalata russa, perfino l'Alitalia. cosa! *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP).* Viviamo in un Paese che, dal punto di vista della salvaguardia e della conservazione dei nostri preziosi beni ambientali e innumerevoli beni culturali, Mongiello).* Mentre il Veneto subisce una delle peggiori alluvioni della storia, con perdite di vite umane, migliaia di sfollati, enormi danni, perfino 150.000 capi di bestiame perduti,

significativa eccezione, quella del suo predecessore. Ieri in quest'Aula il senatore Rutelli ha riconosciuto come, quanto e perché sia ingiusto e ingeneroso

non attuale, ma storica - scarsità di risorse per i beni culturali. Pompei - scrive Bruno Zanardi - non va trattata come una romantica rovina, ma come una città vera e propria, le cui migliaia di case hanno bisogno di tetti, finestre, porte, grondaie e sistemi di smaltimento e canalizzazione delle acque. Una città nella quale vi sono centinaia di edifici in pericolo, abbandonati da anni al degrado perché non esiste più da molto tempo la squadra addetta alla manutenzione ordinaria. È questa la ragione che portò lo scorso anno l'Esecutivo a decidere il commissariamento. Il degrado di Pompei era stato per anni denunciato dai giornali campani, ma quello che succede a Napoli non interessa al resto del mondo. Ci vollero molti interventi per convincere la grande stampa nazionale ad occuparsi del degrado di Pompei.

per accelerare l'opera di conservazione e superare il lungo elenco di provvedimenti e superare il lungo elenco di provvedimenti (notifiche, vincoli, divieti) che limita ogni azione della

essendo impossibilitato a spenderli per l'elevato numero di adempimenti (11, per la precisione) che paralizzano ogni iniziativa. Negli ultimi anni invece - lo dichiara il direttore generale per l'archeologia, professor Stefano De Caro - l'area degli scavi, messa in sicurezza, è più che raddoppiata nell'ambito nell'ambito dei monitoraggi e dei collaudi eseguiti nel 2005. In questo momento a Pompei vi sono 70 cantieri che si occupano del consolidamento degli antichi edifici. Per quanto riguarda la *domus* dei gladiatori, bisogna risalire indietro nel tempo per capire le cause che hanno provocato il disastro: bombardata durante la guerra, fu ristrutturata dal Genio civile negli anni '50 con materiali incongrui e incompatibili. Il solaio, poggiante su mura millenarie, fu realizzato in pesante cemento armato e non con travi di legno, come ai tempi dei romani. Proprio accanto a una delle pareti vi è un terrapieno, costituito in gran parte da cenere e lapilli, che assorbe acqua come una spugna. Le fortissime piogge di questo autunno - ve ne siete per caso accorti? - hanno appesantito il terreno, aggravando infiltrazioni e provocando il crollo di una parete e conseguentemente il crollo dell'edificio sotto il peso del solaio

solamente il restauro eseguito negli anni '50. Non si può quindi sostenere che il ministro Bondi abbia governato male l'esistente. Semmai bisogna risalire alle soprintendenze archeologiche di Amedeo Maiuri, del suo successore Baldo Conticello, e per 15 anni di Giovanni Guzzo. segnalò un imminente pericolo specificatamente per la *domus* o mise mano a strutturali restauri conservativi. Ora la colpa sarebbe del ministro Bondi e del commissario Marcello Fiori che, in due anni, si sono prodigati per fronteggiare centinaia di emergenze. Emergenze che, fino ad oggi, sono state sono state considerate addirittura inesistenti dalla Corte dei conti. Non è un caso, questo, di pregiudizio *ad personam* o, peggio, un pretesto per una mozione di sfiducia individuale, strategicamente presentata in clima di guerriglia parlamentare? Forse qualcuno ricorderà i crolli

accadimenti sia stata avanzata una mozione di sfiducia, come avviene oggi nel caso del ministro Bondi, nei confronti dei titolari dei Beni culturali, si chiamassero Paolucci, Veltroni, Melandri, Urbani

Signor Ministro, non chiedo le sue dimissioni a titolo personale. La mia cultura, il senso dello Stato, delle istituzioni e delle responsabilità non mi consentirebbero nessun tipo di speculazione. Però, mentre non credo che lei abbia una responsabilità personale, ritengo piuttosto che vi sia una responsabilità collettiva del suo Governo. La responsabilità è sempre del Governo e non può essere mai della singola persona quando esiste una gestione che, quantomeno, dovrebbe essere collegiale. Ritengo però, signor Ministro, che la questione dei beni culturali debba essere considerata come mai è stato fatto, né dal Governo Berlusconi né da quelli precedenti, una priorità strategica del nostro Paese. E se è tale, la questione dei beni culturali va tenuta in considerazione diversamente, ha bisogno di finanziamenti, e ha bisogno di non essere considerata sempre in termini di cultura dell'emergenza, vale a dire soltanto ricorrendo alla Protezione civile, ma attraverso interventi strutturali. Una programmazione per la tutela che manca da troppo tempo. Così come ritengo altrettanto giusto che, come esiste presso il Ministero dell'economia un fondo che viene automaticamente rifinanziato per i beni di culto, vi sia la possibilità di finanziare e rifinanziare costantemente (perché ce n'è assoluto bisogno)

si tratta di dieci banche) hanno convinto 350.000 risparmiatori a sottoscrivere azioni ENEL Green Power a un prezzo

Signora Presidente, si tratta di questioni che riguardano il risparmio degli italiani e della povera gente. Voglio ricordare che nel prospetto informativo approvato dalla CONSOB

nelle fauci di questi istituti di credito che convincono, con la pubblicità e con le campagne di stampa, che le azioni sono un affare, ed invece non lo sono,

le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie del pubblico impiego della scuola, secondo quanto previsto dalla legge Bassanini-D'Antona della fine degli anni '90. Queste elezioni non si faranno il ministro Brunetta non le ha indette e non ha neanche modificato la legge o fatto una proposta di rinvio. È un fatto di una gravità eccezionale. Tre milioni di persone sono state scippate del diritto di voto.

in questo momento si sta distruggendo l'impianto del suo lavoro. Tale vicenda ha anche alcuni effetti pratici sul lavoro delle nostre Commissioni. suddetta legge, si prevedeva che i sindacati che non raggiungevano un certo *quorum* non erano rappresentativi e non avevano dunque diritti sindacali, distacchi

si ritiene siano necessari fino a 160 milioni di euro per dismettere le munizioni in nostro possesso e contribuire anche ad una serie di iniziative volte a dare un aiuto ai Paesi vittime dell'utilizzo di queste bombe.

ne va ancora una volta della nostra reputazione all'interno delle organizzazioni multilaterali, sia perché si sta parlando di aiuti concreti nei confronti di popolazioni civili che hanno subito da anni l'uso di queste bombe. *(Applausi